Presidente, nell'apprezzare la diligenza dei colleghi che sono presenti dall'inizio della seduta, non chiediamo la verifica del numero legale.

il senatore Cossutta fa parte di un passato ben preciso, forse è l'ultimo comunista che ha ancora preso i rubli dall'Unione Sovietica.

corone e marchi che sono serviti, forse provenendo dalla stessa fonte, per armare quella mano che, qualche centinaio di metri da qui, ha sparato al Pontefice. Era la stessa parte.

quella legge Biagi che, tra l'altro, anche molti di voi riconoscono come positiva)

persone si sono rivolti; quindi saranno 250.000 o 300.000. Chi paga non interessa, giustamente, alla sinistra. Chi pensa ancora che ci sia una lotta di classe in Italia, in cui questo è il proletariato e gli altri sono i nemici di classe, dimentica - colleghi, va bene che è mattina il manifesto «Anche i ricchi piangono»? Ma è questo che vogliono: che i ricchi piangano e che paghino! E i ricchi, nella coerente concezione della sinistra

senatore Rotondi, credo

Non nostalgici della Democrazia Cristiana, quale io sono, ma economisti e studiosi hanno persino riabilitato alcune pratiche

successive ha animato un dibattito su modalità diverse di strutturazione del rapporto di lavoro, non solo nell'area privata ma anche in quella pubblica. Quindi, il tipo di contratto comunemente definito precario corrisponde ad una riforma della pubblica amministrazione, che risente dell'iniezione liberale intervenuta nel pensiero politico italiano nell'ultimo decennio. decennio. L'iniziativa del senatore D'Amico corrisponde non dico ad un ripensamento, ma probabilmente a una valutazione in corso d'opera di quanto avvenuto. Figure professionali, richiamate ad un ruolo sul presupposto non di una precarietà ma di un rapporto di tipo liberale (non stabile o all'antica, per intenderci), probabilmente invecchiando accusano un dato di precarietà che induce a una riflessione. Questo, però, non è un tema che si possa affrontare in finanziaria. Se mi è permesso rispetto al senatore D'Amico io vedo un ribaltamento di ragione sociale, perché questo emendamento lo si poteva attendere dai banchi della Democrazia Cristiana o delle due obbedienze del Partito Comunista, ossia dalle forze politiche che destra e sinistra

perché siamo di fronte ad un emendamento che prenota un disagio ed un'aspettativa sociale e che è destinato a diventare una mina vagante, rombante e forse esplodente in settori vitali della pubblica amministrazione. E siccome, signor Presidente,

il senatore D'Amico contro i collaboratori dei politici esclusi da ogni tipo di stabilizzazione, giustamente, così ha detto, perché sono i collaboratori della casta, quindi sono la castina, ed è giusto che muoiano nella precarietà: loro, poveri *travet* di segreterie ministeriali, portaborse di Sottosegretari schifosi, vadano all'inferno. Signor Presidente, nella sua segreteria particolare, in quelle del presidente Marini e dei Segretari di Presidenza, tra i collaboratori dei Gruppi quanti ce ne sono in quest'Aula, ci sono dei precari o no? o no dei signori e delle signore che ci scambiamo ad ogni legislatura con il contrattino, che sono venuti qui a vent'anni, affascinati forse anche loro dal film «Il portaborse» che presagiva la castina, che ci palleggiamo da due o tre legislature, che magari nel frattempo hanno messo su famiglia? Siete bravi legislatori secondo voi se fate le leggi sui precari degli altri e a vivere, voi, di lavoro istituzionale sul lavoro precario e, diciamo la verità, qualche volta anche nero? Come vedete, i problemi sono abbastanza complessi e se li affrontiamo, anziché con un ripensamento di carattere culturale, a colpi di emendamenti clientelari non solo affondiamo la finanziaria, ma anche quel tanto di passi avanti che in questa materia una cultura autenticamente liberale ha potuto fare.

Province come Benevento, Potenza, Matera ed Agrigento. Vorrei anche comunicare che i senatori Buccico, Viceconte, Taddei e Gentile aggiungono la firma a questo emendamento.

Presidente, faccio rilevare che comunque ci sarebbero problemi di copertura, nel senso che sia la prima parte, sia la seconda

che l'approvazione di una norma come questa rischierebbe di mettere in discussione il lavoro di un anno, considerando comunque che il problema di garantire un minimo di presenza dello Stato nelle Province più più in difficoltà e di minore densità demografica è effettivo, inviterei il senatore Izzo a presentare un ordine del giorno in tal senso, affinché all'interno del procedimento in atto il Governo valuti, compatibilmente con le risorse finanziarie, cosa è possibile fare e cosa no. Non so se il Governo

sulla riorganizzazione degli uffici, lo schema di Regolamento che è stato approvato dalla 1a Commissione, condizionato al fatto che non derivino nuovi ed ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato. Se voi prevedete una spesa di 4 milioni di euro per il 2008 e di 9 milioni di euro per il 2009, potete benissimo riorganizzare gli uffici; fermo rimane l'orientamento del Governo,

2006 n. 296 assicura in ogni caso la permanenza della Direzione territoriale dell'economia e delle finanze e della Ragioneria territoriale dello Stato nelle Province con una popolazione superiore a 250.000 abitanti»,

Il Ministero dell'economia e delle finanze, in seguito all'approvazione delle norme contenute nella finanziaria, è stato oggetto di una proposta di profonda revisione e ristrutturazione; da un lato è adesso in discussione nelle competenti Commissioni una bozza di nuovo Regolamento, dall'altro vi è un piano di ristrutturazione che tende a contemperare sia gli obiettivi che sono stati ora ricordati dal senatore Izzo, sia il miglioramento dell'efficienza, tenuto conto del tipo e della quantità di attività che viene svolta nelle varie sedi periferiche. Se ho compreso bene la proposta,

di inserire come raccomandazione una formulazione di questo tipo e - auspicherei - anche con un riferimento più generale alla presenza dello Stato e meno puntualmente riferita al Ministero dell'economia e delle finanze, a questo punto posso esprimere un parere favorevole. Mi pare che le cose siano chiare: la proposta non è stata accolta. Se lei, senatore Izzo, non accetta la trasformazione in ordine del giorno dobbiamo votare prima Presidente, la risposta del Governo è assolutamente evasiva e, credo, anche offensiva per quelle realtà territoriali. Che significa la presenza dello Stato? Noi stiamo parlando degli uffici finanziari, non già della prefettura o della questura: questa l'abbiamo già, signor rappresentate del Governo. Che modo di rispondere è questo? Mi sento assolutamente depresso rispetto a questa risposta; vuol dire che sono insoddisfatto e chiedo di votare l'emendamento, così come avevo già preannunciato, per parti separate: primo comma e secondo comma. Il centro‑sinistra Il centro‑sinistra si assume la responsabilità di cancellare gli uffici finanziari nelle realtà più piccole del Paese. Non riesco a capire che sensibilità ha questa sinistra rispetto ai problemi seri che poniamo all'attenzione del Parlamento. bene, c'è una richiesta del senatore Izzo e c'è un'opposizione da parte del relatore alla votazione per parti separate. Devo, pertanto, mettere prima in votazione la possibilità di votare per parti separate. Procederemo con il sistema elettronico senza registrazione dei nomi, così è più chiaro.

la discussione su questo articolo è sembrata un po' surreale. È stato detto che è un articolo di vecchi e nuovi comunisti e, se così fosse,

l'idea di precarizzazione per una più alta idea della civiltà del lavoro; si sono misurate lì diverse culture politiche, e vorrei ricordare qui Guido Miglioli, che è tra i fondatori del Partito Popolare con Sturzo, espulso dal partito per la sua amicizia con Gramsci. Dopo molti anni e anche molte sconfitte, culture politiche diverse affrontano un tema che riguarda un'intera generazione,

È stato detto che questa finanziaria è un incubo. No: è un incubo il contratto temporaneo, interinale, stagionale. È un incubo il contratto di inserimento, la chiamata Co.co.co, la prestazione d'opera occasionale. Questo è l'incubo, quello che vive un'intera generazione. Gli stessi dati, usciti l'altro ieri, del Ministero del lavoro segnano questa condizione: 2,7 milioni di lavoratori, soprattutto donne, ed in particolare ad alta scolarizzazione, sono nella condizione di precarietà. Altro che mammoni o bamboccioni! L'unico ammortizzatore sociale per quella condizione resta spesso la famiglia. I dati I dati del Ministero del lavoro mostrano che spendiamo 2,4 miliardi di euro per incentivare l'apprendistato,

Sarà capitato anche a voi di arrivare ad un distributore automatico e, non sapendo come funziona, di impiegare 10 minuti per capirlo. Ebbene, quando vedete un giovane che magari sta lì a fare quel certo lavoro dovete sapere che, appunto, è un apprendista e guadagna la metà di quello che guadagnerebbe un operaio in quella stessa condizione. È stato detto che questa è un'operazione clientelare. Altro che clientela! Questa è un'operazione che ricostruisce una possibilità, parla ad una condizione sociale della lotta contro la precarietà. io penso, un motivo valido per far parte di una coalizione pensare che dalla scorsa finanziaria sulle questioni che riguardano la scuola e la condizione di precariato con questo si dà una risposta a centinaia di migliaia di lavoratori che, come ricordava lucidamente e con forza il senatore D'Amico, spesso vivono nella loro condizione di un controllo sociale proprio per la loro condizione di precarietà: attraverso questo articolo si offre loro, appunto, la È stato qui ricordato come questo articolo potesse rammentare la legge 1° giugno 1977, (ministro del lavoro Tina Anselmi), ed io ho pensato tra di me: magari fosse una lotta alla disoccupazione, come quella la legge n. 285, che sottrasse, appunto, tanti giovani dalla condizione di ricatto e di controllo sociale nella loro ricerca del lavoro. Per questo noi non solo votiamo con convinzione questo articolo, ma pensiamo che sia un segno preciso, appunto, diretto a quella generazione per farla uscire dalla condizione di precarietà.

uscire dalla sua condizione di precarietà nemmeno attraverso questo articolo, perché - appunto - assunto nella pubblica amministrazione attraverso altri meccanismi. Ma ci sono molti molti altri lavoratori e lavoratrici che danno servizi alle persone nei pubblici uffici, nelle amministrazioni locali, nelle aziende sanitarie locali. pensiamo si possa rispondere e segnare un'altra idea di civiltà del lavoro e della condizione nel nostro Paese.

oltremodo interessante. Vorrei anche ricordare ai senatori che interverranno dopo il senatore Zuccherini, che ieri la Presidenza ha assunto la decisione di dare cinque minuti

di equità sociale (sarebbe meglio dire di risarcimento sociale) sia diventata, nel cinismo un po' disinvolto di una certa politica, un'operazione clientelare. Al contrario del senatore Rotondi, credo che il clientelismo, che pure ha segnato tanti anni della storia dell'Italia, abbia prodotto tante devastazioni sociali, abbia prodotto addirittura delle differenze fra aree del Paese e credo che ancora oggi in parte lo stiamo pagando, anzi ne sono certa. Non sono d'accordo, quindi, su quella valutazione che faceva. Considero questo articolo davvero molto importante. Sono due anni che ci battiamo per arrivare a questo risultato; questa volta, con l'aiuto di tutta la maggioranza, in un clima fortemente solidale, fortemente unitario, siamo riusciti ad arrivare alla scrittura di una norma garantista, rigorosa, severa, ma - come dicevo all'inizio - di grande, dovuto risarcimento sociale alle tante lavoratrici e ai tanti lavoratori che sono impiegati nel pubblico impiego. Pensate, colleghi, alcuni da 12-13 anni 12-13 anni sono precari, fanno esattamente lo stesso lavoro dei loro colleghi, prendono la stessa paga, solo che il contratto viene chiamato Co.co.pro, a termine, LSU: insomma, una situazione di ingiustizia sociale spaventosa. Da questa norma restano fuori - e me ne dispiace molto, è per questo che voglio dirlo - i lavoratori con contratto interinale, interinale, perché sul piano giuridico il loro contratto è con una agenzia privata. Pensate che questi lavoratori costano allo Stato circa il 30 per cento in più degli altri lavoratori, che è la quota che viene data all'agenzia interinale.

là. Ho ascoltato il senatore Angius che, in uno intervento molto severo, a un certo punto ha detto che il precariato non esiste solo nella pubblica amministrazione. Lei ha ragione, senatore Angius, il precariato che esiste nei settori privati è anche più drammatico di questo. Porto un esempio vero, non inventato: nella FIAT, la nostra più grande impresa italiana,

la FIAT ha deciso di assumere dei lavoratori precari che lavorano il venerdì, il sabato, la domenica e il lunedì, che svolgono esattamente lo stesso lavoro degli altri, prendono la metà della paga e non hanno alcun diritto. Ma scuote la coscienza dell'Aula una condizione operaia di questo tipo? Noi qui, senatore Angius, segniamo un'inversione di tendenza, credo. Sarà molto complicato nel settore privato, ma lei ha ragione, dobbiamo metterci le mani, dobbiamo creare un Paese più giusto, più equo, più solidale.

e soprattutto alla persona del sottosegretario Sartor, che ci ha aiutato con grande sapere e con grande solidarietà, e ai senatori Legnini e Morando, che pochi stiamo ringraziando in quest'Aula

mi associo sinceramente all'apprezzamento per il lavoro svolto dai colleghi: senza ironia, so che le finanziarie sono sempre un grosso sforzo. sforzo. Questo articolo è probabilmente il più importante di questa finanziaria, perché assume un grande significato sostanziale, ma anche politico, per capire dove sta l'asse di questa coalizione. Intanto abbiamo assistito, tra ieri

Allora, è chiaro che ha vinto, legittimamente, per le sue idee, la parte socialista massimalista di questa coalizione.

Diceva: «Una grande debolezza del sistema Italia è il peso della burocrazia sulle attività economiche. Questo peso non è più sostenibile!»; affermava che bisogna rendere competitivo il Paese e che non è più ammissibile uno Stato che sottrae risorse alle attività economiche». Ebbene, sull'onda di queste dichiarazioni la nostra Bibbia nazionale, il «Corrierone» fa fa questa dichiarazione per bocca del suo direttore Paolo Mieli: votate Prodi, così avremo un Paese più moderno, un Paese più competitivo. Prodi vince le elezioni su queste promesse. Vi è addirittura chi, sempre nel "Corrierone", si avventura a dire: licenziamo i fannulloni dalla pubblica amministrazione;

Vince l'ala massimalista di questa coalizione e Prodi fa una scelta precisa: butta nel cestino tutte le

non sono stati in grado di calare nella realtà umana l'utopia dell'uguaglianza di tutti, della mancanza della proprietà privata: senza proprietà privata, con il mito dell'uguaglianza, nessuno produce più nulla. Vorrei ricordare che il Muro di Berlino è stato buttato giù dai comunisti e non dagli occidentali. Questo forse dovrebbe insegnarci

anziché vantarsi di avere stabilizzato altri 500 precari *motu proprio* della Polizia penitenziaria, si accorgerebbe che abbiamo la Polizia penitenziaria più pletorica del mondo: abbiamo un agente per ogni detenuto. In tutto il mondo ci batte soltanto l'Islanda, che ha 30 detenuti e 36 agenti. Noi abbiamo 45.000 agenti per 44.500 detenuti. Eppure ne vogliono assumere ancora! Ma voi pensate che con un sistema di questo genere si possa essere competitivi, che

la maggioranza dovrebbe contenere al massimo i tempi e, quindi, chiedo un po' di pazienza anche ai miei colleghi.

Nella finanziaria dello scorso anno, abbiamo approvato una norma che, in linea di principio, chiedeva la riduzione della spesa del personale per le amministrazioni locali sottoposte al rispetto del Patto di stabilità.

In questo senso, invece, i commi 30 e 31, che abbiamo introdotto in Commissione, garantiscono agli enti locali la possibilità di assumere personale in deroga al principio della riduzione della spesa, motivandolo in modo molto preciso e dettagliato, ma accompagnando questa possibilità di deroga a dei paletti, a delle condizioni che vanno nella direzione di premiare i Comuni virtuosi. Sono condizioni che entrano nel merito, che chiedono, oltre al rispetto del Patto di stabilità,

una norma che limita in maniera drastica la possibilità per le amministrazioni pubbliche di utilizzare nel futuro gli strumenti delle assunzioni flessibili, che hanno creato nel tempo abusi, precari e clientele, e l'emendamento approvato evita di fatto la sanatoria, condizionando le assunzioni a concorsi e selezioni.

proprio nelle Regioni governate dal centro-destra. È della scorsa settimana un botta e risposta, in soli due giorni, del consiglio regionale del Veneto, nei confronti dell'assessore alla sanità, che è stata messa in minoranza da tutto il consiglio regionale, il quale non da tutto il consiglio regionale, il quale non si è accontentato di una mozione ma, addirittura, in due soli giorni ha approvato una legge, che impone alla giunta regionale di stabilizzare

va affrontato all'interno della questione più generale della riforma della pubblica amministrazione; è di primaria importanza razionalizzarla e saper guardare dentro alla macchina, per capire perché le organizzazioni pubbliche non funzionano nel migliore dei modi. Questa è una riforma che costituisce una sfida sia per la maggioranza che per l'opposizione, come dimostra la circostanza che l'opposizione ha censurato le norme sulle stabilizzazioni del personale come lassiste, ma poi esulta quando passano con il suo voto emendamenti che vanno nella direzione contraria al rigore, come è successo anche questa mattina. Signor Presidente, nella mia città, quando ero adolescente, c'era un signore, che mi ha sempre affascinato, che aveva tre carte e faceva uno strano gioco: «Qui c'è, qui non c'è», e la carta non si trovava mai. Devo dire, sinceramente, che la discussione su questo articolo mi ha fatto tornare in mente quella situazione dell'infanzia; è così che si sta comportando la maggioranza.

Si è detto che si voleva ripristinare l'obbligo del concorso per l'accesso alla pubblica amministrazione, così come prevede l'articolo 97 della Costituzione, che parla per l'appunto di concorso; l'emendamento D'Amico, infatti, in maniera più oscura parla di «procedure selettive di natura concorsuale o previste da norme di legge». Qui si è fermato ieri sera il senatore D'Amico, io ho interrotto invitandolo ad andare avanti nella lettura. L'ho fatto con irruenza, e me ne scuso, anche se gli ricordo che le interruzioni, quando sono un'interlocuzione, appartengono alla nobiltà della tradizione parlamentare.

*escamotage* per evitare, appunto, la regola del concorso. La carta si è fatta prima vedere e poi si è nascosta. Il secondo criterio che l'emendamento D'Amico ha voluto introdurre

potranno essere stabilizzati con normativa da fissare entro marzo 2008. Ancora una volta, la carta prima viene fatta vedere e poi viene nascosta. Concordo con il senatore D'Amico che

di «riconoscimento, in termini di punteggio, del servizio prestato presso le pubbliche amministrazioni», senza specificare l'ammontare di questo punteggio. Molto probabilmente, avremo concorsi riservati con una quota

stabilizzati, altri 399.000 nutriranno la legittima aspettativa, giuridica e morale, di esserlo. Avremo così una sindacalizzazione del precariato. Abbia il coraggio di mettere in correlazione questa affermazione (perché lei ha parlato di assunzioni clientelari) con la realtà di 75.000 giovani che hanno affrontato un concorso, lo hanno vinto e stanno stanno perdendo il diritto di essere assunti! Spero che la senatrice Palermi conservi ancora un margine d'indignazione da riservare a questi giovani, ai quali lo Stato ha chiesto impegno, tempo, e che poi ha lasciato fuori dalla porta. Signor Presidente, un buon legislatore deve anche saper fare empatia. Cosa faranno oggi faranno oggi un giovane che ha superato un concorso o un genitore che ha affrontato dei sacrifici per portare il figlio a vincere un concorso in maniera regolare,

signor Presidente, stiamo creando l'illusione di combattere il precariato (perché solamente mille precari verranno sistemati) e, insieme, la certezza

lo si vorrebbe fare attraverso una bollinatura liberal-democratica: ebbene, signor Presidente, non lo consentiamo. Riconosciamo al senatore D'Amico che il suo è stato un tentativo suo è stato un tentativo generoso che però ha come presupposto il fatto che questo articolo debba essere per forza approvato. Ebbene, c'è un modo per sottrarsi a tutto ciò, per affermare veramente dei princìpi liberali e di democrazia, ed è quello di bocciare questo articolo. Non è essenziale a questa finanziaria e sarebbe un segnale forte di civiltà che noi daremmo al Paese.

di tener conto in qualche modo di questo dramma che si vive attualmente nel nostro Paese, in presenza di un periodo certamente non felice, quindi con le speranze e le aspettative che noi dobbiamo

L'evidenza di una sistemazione così, pura e semplice, *ad* *libitum*, di chi comanda in questo momento nel Governo era chiara e ha preoccupato tantissimi di noi, come è emerso negli interventi giustissimi che sono stati svolti. Voglio ringraziare il senatore D'Amico, il quale ha compreso che la strada indicata dagli emendamenti aggiuntivi per la sistemazione dei precari nella pubblica amministrazione non poteva avere una prospettiva di realizzazione perché, dai calcoli che tutti abbiamo fatto, risulta che, anche con l'aumento

di non aggravare la situazione facendo delle promesse che non possiamo mantenere; ciò evidentemente va al di là dell'attuale Governo, domani qualunque Governo si troverà di fronte a questo tema, quindi è bene che si fissino in questo momento

sono tutti *escamotages* che sono stati adottati negli ultimi tempi per superare l'unica regola per entrare nella pubblica amministrazione, la regola aurea che noi dobbiamo difendere se vogliamo difendere il merito: che si entra nella pubblica amministrazione mediante procedure concorsuali pubbliche, perché questo è il cardine della meritocrazia e della scelta che si fa per la pubblica amministrazione. Per questi motivi, non essendoci né i soldi per sistemare gli aventi dirittoné i criteri che legittimano l'assunzione nella pubblica amministrazione con il merito, voteremo contro - mi dispiace - questo emendamento

pubblica amministrazione e del personale nel nostro Paese, siano strategici per il futuro della nostra comunità.

le nostre imprese. Quello che avviene sul territorio nazionale è singolare: il Paese rischia di essere sopraffatto dalla criminalità organizzata,

quotidianamente in tal senso. Questo non vale soltanto per le forze dell'ordine, ma anche per il settore della giustizia (uomini che hanno un vero senso dello Stato, uomini e donne che difendono e promuovono politiche serie di giustizia, senza invadere il campo degli altri poteri nel nostro Paese). Con questa consapevolezza, signor Presidente, vogliamo mettere l'accento anche su quello che riteniamo insufficiente in questo articolo e nell'architrave generale della finanziaria.

della sicurezza fatto per una lotta politica interna, dove l'interesse generale è stato messo da parte perché è prevalso l'interesse di coalizione, di una sinistra radicale che anche su questi temi è riuscita a sopraffare quell'utopia del Partito democratico appena nato che sulla sicurezza poteva e voleva dire qualcosa. Questo ci sembra il punto politico. Ma tutto questo, signor Presidente, onorevoli colleghi, non deve farci riflettere perché in ogni scelta politica della finanziaria e, in generale, in ogni scelta amministrativa dobbiamo sempre ricordare che vi è una persona in carne ed ossa; una persona che aspetta dal Parlamento, dalla buona politica che non arriva, una risposta significativa. Con le nostre iniziative, con tutto quello che abbiamo voluto dire per evitare di far diventare questa Aula uno scontro tra tifosi, abbiamo voluto mettere la nostra capacità ed il nostro buonsenso al servizio della finanziaria, proponendo emendamenti non ostruzionistici. Ma noi dell'UDC per primi abbiamo voluto dare abbiamo voluto dare il nostro contributo sui temi della sicurezza e della pubblica amministrazione, ma in generale, signor Presidente, su tre grandi temi,

ad una qualità del nostro ordinamento che doveva marciare in un certo senso. Dall'altra parte, anche sulla sicurezza, con gli emendamenti che abbiamo presentato (io stesso ho presentato un emendamento che discuteremo nei prossimi giorni in questa Aula

un'unità nazionale, dove persone che la pensano allo stesso modo possano ritrovare logiche di Governo, logiche volte a fare il bene del Paese e l'interesse generale, che non può essere sottoposto all'interesse particolare dei tifosi, allo scegliere tra bianco e nero. Per concludere, nelle nostre indicazioni abbiamo sottolineato che il territorio, lo diceva il collega Mantovano, collega Mantovano, si controlla anche con il coordinamento delle risorse. Non vogliamo fare degli *spot* pubblicitari, diciamo che le forze dell'ordine devono essere sostenute, dobbiamo prevedere maggiori sostanze, maggiori finanziamenti, ma la capacità di Governo si deve esplicare anche nell'indirizzo di come questi soldi devono essere spesi. Non possiamo, onorevoli colleghi, dare soltanto finanziamenti a pioggia, dobbiamo distinguere tra Carabinieri e forze dell'ordine, e valutare come tali stanziamenti devono essere finalizzati nella sicurezza del territorio. Sui precari, signor Presidente, volevo dire che la riforma della pubblica amministrazione, e concludo, è un fatto serio. Dimentichiamo spesso che tutto questo dibattito rischia di diventare ideologico. Dobbiamo superare questo odioso problema del precariato, lo diceva il collega Quagliariello.

diciamo al Governo, che è il datore di lavoro, di dire chiaramente cosa si vuole da queste persone che lavorano. Non possiamo lasciarle lì senza alcuna indicazione politica e di Governo, dobbiamo dire qual è il nostro obiettivo e su questo l'UDC darà sicuramente il suo contributo.

Signor Presidente, signori del Governo, onorevoli colleghi, vorrei fare una breve dichiarazione di voto favorevole a questo articolo, il quale risponde ad un'esigenza di equità sociale ma anche di ripristino dello Stato di diritto. Con l'approvazione di questo articolo si avvia un processo di cessazione di un fenomeno scandaloso, quello del ricorso in gran

stiamo parlando: di Vigili del fuoco, che in un Paese che attualmente non è ancora in adeguate condizioni per sconfiggere fenomeni di incendio come quelli che si sono verificati questa estate, sono in buona misura dei precari; stiamo parlando dei bidelli delle scuole, senza i quali le scuole non potrebbero funzionare, stiamo parlando quindi di lavori pieni e permanenti nel tempo, per i quali quindi il ricorso al contratto precario è una frode; stiamo parlando di vigili urbani, di centralini del Ministero e così via. È stato uno scandalo durato troppo a lungo che deve cessare, per questo la norma che stiamo per approvare si basa su due principi: il primo è mai più ricorso al precariato nel pubblico impiego, il secondo è avviare un piano graduato nel tempo di progressivo riassorbimento di questi lavoratori precari, purché sia rispettato il principio della procedura selettiva secondo quanto richiede la nostra Costituzione. solo non si fa un favore a nessuno, anche se a volte dovremmo ricordarci che qualche favore alla povera gente lo potremmo anche fare, nel momento in cui si controverte addirittura se sia giusto porre un tetto

del nostro sistema della pubblica amministrazione che è in primo luogo di moralizzazione, perché d'ora in poi ci saranno solo concorsi veri per l'ingresso nella pubblica amministrazione, in secondo luogo di funzionalità del sistema, in terzo luogo di equità sociale. È una proposta certamente di sinistra, ma è anche una proposta liberaldemocratica per chi chiede, nello Stato di dritto, la correttezza di rapporti tra le pubbliche amministrazioni e i loro dipendenti.

Il senatore Castelli è l'ex ministro della giustizia, e per tutti i problemi che lui ha rappresentato in quest'Aula, in questa legislatura ha avuto cinque anni di tempo per risolverli; fatto? Queste sono le domande che mi pongo; si fa della facile demagogia, soprattutto quando si riportano dati sbagliati

in quanto ci sono anche altre questioni che vivono gli stessi agenti: malattie, ferie, eccetera. Lanciare sempre messaggi sbagliati non è utile, il Paese ha bisogno di serietà.

il Movimento politico dei cittadini ha già espresso voto contrario al capitolo sull'ambiente, voto contrario al capitolo che riguarda le guerre e gli armamenti. Il nostro orientamento era quello di esprimerci con voto contrario anche su questo, perché temevamo, date le notizie di stampa, secondo le messo il bastone tra le ruote della politica sui precari, che avvenisse qualcosa di intollerabile anche su questo. Devo ammettere che invece l'intervento del senatore D'Amico, e nel merito il risultato del lavoro della Commissione, sono apprezzabili; condivido tutte le parole del senatore D'Amico e a chi lo accusa di non essere liberista, vorrei ricordare che Keynes era un liberista; dice, per quanto riguarda questa finanziaria e questo articolo, che siamo in presenza di socialismo reale, devo dire che già a me piaceva poco quello, ma se questo fosse socialismo reale, con questa finanziaria mi piacerebbe ancor meno. Qui siamo in presenza, purtroppo, di fenomeni che appartengono al capitalismo reale, non al socialismo reale che non c'è più, mentre il capitalismo c'è. C'è con i milioni di poveri che ci sono nel nostro Paese (anche se li chiamiamo incapienti) e c'è con i giovani incerti sul proprio futuro. Un Governo, sia esso di centro-destra o di centro-sinistra,

costretti a stare in casa perché non hanno sicurezza sul proprio futuro e non hanno risorse adeguate per metter su la propria famiglia. Questo non lo dicono quelli del capitalismo reale; lo dice la Chiesa cattolica, anche se i Teocon se ne dimenticano. Ci sono delle ingiustizie profonde nella società. Quando si parla di criminalità e si lascia un giovane meridionale senza occupazione, in mano a chi lo si mette? Allora, ci sono questioni sociali da affrontare. Purtroppo, con questa finanziaria non le risolviamo, ma la porta resta aperta e noi speriamo che tra ordini del giorno ed emendamenti ci siano maggiori speranze e che il numero dei dei precari nel pubblico, che possano trovare lavoro stabile, possa crescere utilizzando i fondi dormienti. Signor Presidente, come è stato già ricordato negli interventi che mi hanno preceduto, il precariato è davvero un problema sociale molto grave

del fenomeno presente nel nostro Paese. Il problema riguarda milioni di persone che lavorano e soprattutto le donne e i giovani diplomati e laureati. Qui, non c'entra proprio niente la necessaria flessibilità cui, a volte, bisogna ricorrere per far fronte alle esigenze anche della pubblica amministrazione. Qui, sovente si ricorre alla prestazione precaria per far fronte a problemi di costo, utilizzando anche politiche di bassi salari che vanno soprattutto a scapito dell'efficienza e della produttività della pubblica amministrazione; altro che favoritismi e clientelismo. Sono queste le ragioni che ci portano a votare, come Gruppo dell'Ulivo, convintamente a favore dell'articolo 93.

*(AN)*. Signor Presidente, chiedo all'Assemblea e a lei, signor Presidente, di procedere alla votazione dell'articolo 93 per parti separate, distinguendo dall'intero corpo dell'articolo il comma 29 e, se me lo consente, vorrei indicare brevemente le ragioni di questa richiesta.

una spesa di mezzo milione di euro per l'assunzione di 22 educatori professionali da attribuire al sistema penitenziario per la Regione Piemonte. Piemonte. Signor Presidente, è lungi da me l'idea di sollevare una qualsiasi censura sull'iniziativa dei senatori che hanno proposto l'emendamento che poi è stato votato dalla Commissione bilancio. senatori appartenenti alla regione Piemonte che hanno svolto con diligenza e attenzione il loro mandato. Non altrettanto posso dire nei confronti del relatore in Commissione bilancio,

a comprova del fatto che non vi era alcun atteggiamento ostruzionistico da parte dell'opposizione nel corso dell'esame di questa legge finanziaria, ma che vi era il forte reclamo, nel caso specifico, nei confronti proprio del Ministro guardasigilli, perché egli stesse permettendo quanto oggi si verificherà. Si interverrà infatti nel sistema di distribuzione del personale di assistenza alla popolazione detenuta in chiave assolutamente atipica, per la prima volta che io sappia nella nostra storia, con una violazione di più precetti costituzionali, tra cui spiccano il diritto alla parità del trattamento e quello della rieducazione della pena. pena. Signor Presidente, le chiedo scusa se mi dilungo su questo aspetto che ad alcuni potrebbe sembrare secondario, ma io credo che si sta verificando un fatto assai grave: gli educatori che mancano nel nostro sistema penitenziario - ho sotto gli occhi l'aggiornamento al 15 ottobre del Ministero della giustizia - sono 725 unità in tutto il Paese. Non vedo la ragione per cui i

e attenta alle questioni attinenti al sistema di trattamento penitenziario. Chiedo, signor Presidente, che il Ministro guardasigilli si esprima espressamente su tale disposizione, per dire se egli concorda

voto. Vorrei cortesemente chiedere l'attenzione su questo argomento, perché in effetti stiamo parlando di quegli ufficiali in ferma prefissata che che hanno superato i 36 mesi di servizio e, già in base al comma 519 della finanziaria dell'anno scorso, avrebbero dovuto trovare una sistemazione di stabilizzazione.

Grazie, signor Presidente. Purtroppo non solo non si è avuta questa stabilizzazione, pur essendoci un richiamo espresso nel comma 519 della finanziaria dell'anno scorso,

ma anche quest'anno questi ufficiali, che sono circa 1600, vengono ancora una volta non considerati e pertanto non trovano alcuna procedura di stabilizzazione. Rappresentano, tra l'altro, persone che hanno acquisito professionalità: di fatto su di loro c'è stato un investimento, hanno superato i 36 mesi di servizio

rappresentante del Governo di porre attenzione e, qualora non ritenessero opportuno accogliere l'emendamento, atteso già quello che è stato il parere espresso, vorrei chiedere se

ai Corpi di polizia e ai Carabinieri di attingere nelle assunzioni ai soggetti che sono indicati nell'emendamento stesso. Quindi, nel confermare

Vorrei dire anche all'Assemblea che il miglioramento dell'amministrazione pubblica non passa per l'indiscriminato aumento di dipendenti perché averne uno che non fa niente e metterne un altro che non fa niente non cambia nulla, posto che ci siano quelli che non fanno nulla, come afferma il «Corriere della Sera» - ma attraverso il miglioramento dell'efficienza. Credo di essere stato l'unico Ministro,

Il senatore Rossi, molto attento, aveva già individuato il problema tant'è che per scoprire la foglia di fico e vedere cosa ci stava sotto aveva pensato un emendamento che non individuasse soltanto

delle risorse necessarie per la stabilizzazione di uno dei soli precari per il numero dei precari. Si parlava di 30.000 euro per 300.000 precari, 3 per 3 fa 9, ed ecco che si arriva

Non è una provocazione, ma a questo punto diventa una discussione molto più ampia perché la realtà - l'ha detto benissimo il senatore Quagliariello - è che tutto quello che abbiamo fatto è soltanto demagogia e mistificazione, rispetto ad un problema

di prendere seriamente in considerazione le problematiche relative al costo del lavoro nel nostro Paese e, quindi, quelle che

di principio, il posto di lavoro sicuro e tranquillo è un concetto al quale tutti possono aderire; capiamo altrettanto che con l'adozione di questa

meditate: ogni voto non è determinato dalla fretta con cui ci si adegua all'indirizzo, alla scelta e all'indicazione di voto del responsabile del Gruppo che segue e che governa tali indicazioni, ma dobbiamo dedurre che abbiamo compiuto scelte meditate.

a quella che i Gruppi del centro‑destra hanno sostenuto nel corso di questo dibattito. Dal centro‑destra è venuta una critica alla soluzione sostanzialmente riassunta nell'emendamento del

procedure di stabilizzazione che sarebbero considerate dal centro-destra eccessivamente generose nei confronti dei lavoratori precari. La discussione, a mio avviso, ha dimostrato, soprattutto con l'intervento del senatore D'Amico di ieri sera, molto seguito e accompagnato da un larghissimo consenso che, in realtà, questo giudizio è infondato. Vorrei tuttavia far notare che nell'ansia di vedere se si riesce una volta a vincere una votazione, si stanno facendo scelte politiche completamente contraddittorie da parte dei Gruppi dell'opposizione.

quindi non vota - è sempre possibile ed è appena accaduto - però che ci sia l'ansia del centro-destra di mettere in minoranza il centro-sinistra e il Governo su una linea linea del tutto incompatibile con gli indirizzi che il centro-destra mostra di seguire anche nel corso di questa discussione, mi sembra un fenomeno che Vladimir Ilic, una

troppo s'innamora della tattica parlamentare e pensa che la strategia politica possa essere sostituita da iniziative di tatticismo parlamentare prive di costrutto. Questa è la sostanza di quella critica politica.

volto ad impedire il processo di ridimensionamento della presenza dello Stato centrale in periferia.

mi sembra quanto mai ingiustificato. Come Presidente, pur di negarmi la parola, lei ha ricordato l'episodio di ieri.

in contrasto con gli uffici, di ammettere un emendamento che prevede l'invasione delle prerogative degli organi costituzionali e ha motivato l'ammissione di quell'emendamento affermando testualmente che quella ammissibilità lui la decideva sì in contrasto con il Regolamento, ma in base a parametri di valutazione politica. Questo è il ragionamento che è stato svolto dal senatore Morando, presidente della 5a Commissione. Il tutto è rintracciabile nel resoconto n. 165. Presidente, avrebbe il dovere di verificare se le mie affermazioni sono vere o false. false. Se le mie affermazioni sono vere, la Presidenza del Senato ha il dovere di intervenire sul Presidente della Commissione per richiamarlo all'osservanza del Regolamento.

l'opposizione, che è maggioranza elettorale in questa Camera, di cretinismo parlamentare. Ebbene, se c'è una manifestazione di cretinismo e di malafede parlamentare, è quella data dal Presidente della Commissione bilancio.

Volete impedire agli idonei di concorso di accedere ai posti di lavoro che hanno legittimamente conquistato? Allora dovete votare per l'emendamento del senatore Ferrara. Perché se non lo votate, voi siete cretini, in malafede e buffoni!

Va bene la tattica parlamentare, va bene il fatto di cercare di buttare sotto la maggioranza, però non si può votare tutto il votabile. Questo emendamento, consentitemelo, colleghi della Casa delle Libertà, almeno per quanto ci riguarda,

Lo conosco dal 1996 e da allora fino al 2001 ci impartì le sue professorali lezioncine *ex cathedra* con un tono (mi consenta, senatore Morando) veramente insopportabile.

Senatore Morando, per cortesia, lasci perdere queste espressioni che non le fanno onore e credo che il Presidente non le dovrebbe consentire. Se dovessi utilizzare gli stessi suoi metodi le direi che ha portato avanti questa finanziaria dal

finestra"). Mentre la Presidenza esprime il cordoglio a lei e alla città di Matera, di cui è sindaco, ovviamente si attiverà per cercare di portare sollievo in una situazione tanto difficile. **Ripresa della

Come ha confermato in Aula il collega Tecce ieri, la stabilizzazione dei precari, visto che sono già pagati dalla pubblica amministrazione, determina un maggiore onere pari a circa il 30-40 per cento in più rispetto a quello che attualmente già ricevono. Quindi, si stima per 200.000 persone un maggior costo di un miliardo e mezzo. Dall'altro lato, l'articolo approvato e l'emendamento D'Amico appongono solo 20 milioni. Questa non è economia politica, ma ipocrisia politica.

D'altro canto, però, se si stabilizzano, come la stabilizzazione delle aspettative dimostrerà negli anni, 200-300 mila persone, il costo è un miliardo e mezzo o più. L'emendamento Rossi, fatto proprio dal collega Ferrara, mette in evidenza di fronte all'Assemblea la palese ipocrisia che la maggioranza di Governo sta raccontando in Aula e fuori di essa. A nome del collega Caruso, chiudo con una battuta: non ci sentiamo offesi dall'accusa di cretineria politica: se questo bastasse a mandare a casa il Governo Prodi e questa maggioranza sgangherata, ebbene potremmo anche fare i cretini.

la decisione del Presidente del Senato presa all'unanimità dai Capigruppo in modo rigoroso. Non ci esporremo a nessun attacco pretestuoso da parte di altri; non utilizzeremo neanche un secondo in più perché questo fa parte delle regole corrette della vita parlamentare. Mi auguro che tutti i colleghi facciano lo stesso.

Presidente, colleghi dichiaro, il voto contrario del Gruppo di Forza Italia all'articolo 94, nonostante la materia da esso trattata, quella della mobilità del personale delle pubbliche amministrazioni, potrebbe ad una prima lettura indurre a considerazioni positive. Non vi è dubbio infatti che la mobilità è uno strumento straordinariamente necessario per garantire una più corretta distribuzione del personale delle amministrazioni pubbliche, che, com'è noto, oggi è male organizzato, trascurandosi nuovi servizi o servizi di crescente domanda, e, dall'altro lato, rinvenendosi fortissime presenze nel cosiddetto *back office,* cioè nelle funzioni che spesso sono di mero autofunzionamento delle amministrazioni pubbliche, per non dire della pessima distribuzione geografica del loro personale. Ma qui la norma deve essere letta in combinato disposto con i contratti collettivi in corso. Cioè, lo stesso Governo, che qui afferma di voler procedere a programmi intercompartimentali di redistribuzione del personale delle amministrazioni pubbliche, ha realizzato, attraverso l'agenzia a ciò dedicata, l'ARAN, contratti collettivi che impongono la necessità che operazioni di mobilità come queste debbano essere poi imbrigliate nelle maglie della contrattazione; il che equivale ragionevolmente, a paralizzare le operazioni di mobilità, se non a ridurle a pochissime persone. Per non dire ancora del protocollo sottoscritto dal Governo con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, nel quale si è affermata per la prima volta la rinuncia all'autonomo potere di organizzazione del datore di lavoro, riconoscendo alle organizzazioni sindacali poteri di veto nelle materie proprie nelle materie proprie del datore di lavoro, cioè nelle materie appunto di organizzazione, prima fra le quali la mobilità. Quindi, il nostro voto contrario si rivolge ad un provvedimento che non garantisce per nulla il realizzarsi effettivo di grandi processi di mobilità, pur nel quadro delle regole di equipollenza delle funzioni che diversamente dovrebbero essere svolte e della compatibilità con la residenza. Pur in quel contesto questi processi di mobilità potrebbero svolgersi solo se potessero anche avvalersi dell'iniziativa unilaterale delle amministrazioni pubbliche. [**Presidenza del vice presidente

Signor Presidente, cari colleghi, nel 1989 l'Italia perse l'ultima grande occasione per risanare la finanza pubblica. Tre anni dopo, nel 1992, l'Italia si trovò in condizioni difficilissime e perdemmo in cinque giorni 60.000 miliardi di vecchie lire di riserve valutarie. di riserve valutarie. C'è la parte sociale che grida al successo rivendicando di avere, con questa finanziaria, effettuato una redistribuzione sociale del reddito, mi riferisco in particolare al lucido intervento del collega Zuccherini, e c'è dall'altra parte chi dichiara di avere vinto perché ha mantenuto le linee del rigore.

sale al 2,4 per cento con la maggiore spesa approvata dalla Commissione, sale al 2,7 per cento con le maggiori spese decise in quest'Aula, con la grande incognita del costo della stabilizzazione dei precari. Nel frattempo, la crescita economica rallenta e automaticamente rischieremo di sfiorare pericolosamente, l'anno prossimo, il 3 per cento del rapporto *deficit*-PIL, altro che redistribuzione sociale del reddito, altro che rigore della finanza pubblica! Così, come dopo il 1992 - quell'arco di tempo perso, quell'occasione mancata del 1989, con la caduta del Muro di Berlino, dieci anni ci sono voluti per ricostruire un minimo di credibilità, durante i quali chi ha più pagato è proprio la povera gente - il risultato è che non vince è che non vince l'ala sociale, con 81 centesimi alle pensioni minime e 41 centesimi agli incapienti, non vince l'ala rigorista liberal-democratica, con un *deficit* che tende pericolosamente al 3 per cento, nel momento in cui la crescita rallenta. La verità, cari amici della sinistra sociale, è che voi avete votato, dietro queste foglie di fico, una redistribuzione pesante a favore dei capitalisti senza capitali e dei capitalisti con i capitali dei soldi dei tartassati italiani. Concludo con due esempi. Avete introdotto una riforma IRE che sgrava di un miliardo le grandi imprese e le grandi banche e fa pagare 2 miliardi in più alle piccole e medie imprese, e lo sapete voi per primi. Avete rifiutato di prorogare al 2008 quella miseria di 41 centesimi giornalieri agli incapienti, nello stesso istante, negli stessi giorni, in quest'Aula. In realtà, perde l'ala sociale, perde l'ala liberaldemocratica dentro la maggioranza, purtroppo perde l'intero Paese. *(Applausi dal

Ovviamente si tratta di una specificità relativa agli ordinamenti, alle carriere, ai contenuti del rapporto di impiego e alla tutela pensionistica e previdenziale. Si tratta, quindi, del riconoscimento di una specificità vera non soltanto enunciata, com'è accaduto da parte di questo Governo quando abbiamo avuto modo di esaminare il Documento di programmazione economico-finanziaria che dava disponibilità a questo riconoscimento, ma che in sostanza nei fatti non è andato avanti su questa linea. difendere le Forze armate e di polizia in questo momento significa difendere la politica estera di un Paese che sulle Forze armate e sul lavoro dei nostri militari sta tutelando la propria immagine internazionale in seno ai grandi consessi internazionali in cui siamo rappresentati proprio per forza delle nostre missioni di pace. Difendere le Forze armate significa difendere gli uomini in divisa - che spesso, poiché monoreddito, sono al di sotto della soglia di povertà che tutelano la sicurezza dei cittadini e che oggi sono privi di ogni cosa, dai carburanti per gli automezzi alla possibilità di guardare ad un futuro migliore, alla certezza di avere strumenti per contrastare la criminalità sia all'interno che all'esterno del Paese. A questi uomini vengono richiesti compiti importanti, fino all'estremo sacrificio della vita. Per questi uomini si sprecano poche parole e, a stare agli interventi della maggioranza, il programma dell'Unione addirittura, quando parla di spese militari, genericamente si rivolge a una riduzione di spesa che va sempre a infliggersi sul capitolo dell'esercizio che garantisce la manutenzione dei mezzi, il funzionamento dello strumento militare, la capacità di addestrare meglio il personale e cose di questo tipo, che appartengono sì alla sicurezza, ma alla sicurezza di questi cittadini in divisa nei confronti dei quali questo Parlamento e quest'Aula hanno bisogno di dedicare uno scatto d'orgoglio. Chiedo che questo scatto d'orgoglio - che non è un fatto di parte perché spesso in Commissione difesa anche i colleghi dell'Unione hanno voluto far sentire la propria solidarietà presentando emendamenti similari emendamenti similari - si levi da quest'Aula attraverso il voto di questo emendamento che ho presentato insieme al collega Giulio Marini e che questa volta è un po' solitario, perché anche alcuni emendamenti dello stesso tenore, presentati dai colleghi dell'Unione, sono stati respinti. Allora, quanto avete scritto, signori del Governo, nel DPEF era un'enunciazione di principio o era la volontà reale di dare agli uomini in divisa un segnale forte e condiviso? È questo l'appello che faccio: diamo un segnale forte e condiviso per le Forze armate, le Forze di polizia, gli uomini in divisa che in questo Paese tutelano tutti noi e che consentono a voi, signori del Governo, di esplicitare una politica estera degna di questo nome e che oggi si gioca sulla divisa e sulle nostre missioni di pace.

sia in questa legge finanziaria che nella precedente é stata riconosciuta una particolare attenzione destinando delle risorse a fronte del tema della specificità. Quindi, non si tratta assolutamente di negare l'importanza del fenomeno che è stato illustrato in precedenza; si tratta di trovare un giusto punto di equilibrio che sia coerente anche con il complesso degli interventi che vengono proposti e, per quanto riguarda le modifiche di tipo ordinamentale, queste saranno tenute in debito conto via via che si

il senatore Formisano e altri avevano presentato analogo emendamento e quindi speravamo in quello spirito che il presidente Morando ha enunciato poc'anzi.

Signor Presidente, vorrei dire che io e i colleghi Ramponi, Baldassarri, Berselli e Saia abbiamo presentato un emendamento con il quale si specifica la necessità di disciplinare, mediante l'attivazione di apposite procedure previste dallo stesso decreto legislativo n. 195 del 1995 le funzioni svolte per la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica.

considerando anche le argomentazioni svolte dal sottosegretario Sartor. L'emendamento 95.1 pone un problema complesso, che esiste; peraltro la specificità

riguarda i rinnovi della contrattazione per il pubblico impiego e, nell'ambito di questo articolo 95, il comma 4 - lo sottolineava prima il relatore introduce, più che delle risorse, dei limiti all'utilizzabilità delle risorse per la cosiddetta specificità. Vorrei fare una brevissima premessa

con due rinnovi e due code contrattuali, le Forze di polizia hanno ottenuto, in media, a testa un aumento complessivo di 410 euro lordi, che a mio avviso sono insufficienti: però, con quei chiari di luna e in assenza di extra-gettito, probabilmente non si poteva fare di più. In questa legislatura,

vi è stato, con un anno e mezzo di ritardo, il rinnovo del contratto delle Forze di polizia e delle Forze armate, che è consistito in una parte normativa e in una parte economica, che ha riconosciuto in termini non di arretrati, ma di tutto ciò che era maturato dal primo gennaio 2006, semplicemente un *forfait* e, in termini aggiuntivi, le cifre sono assolutamente simboliche. La riprova di tutto questo sta nella rubrica dell'articolo 95 che riporta: «Integrazione risorse rinnovi contrattuali, biennio 2006‑2007». Quindi, il testo della finanziaria ammette che il rinnovo contrattuale per le Forze di polizia e le Forze armate nel biennio che sta per concludersi è avvenuto senza risorse, se pudicamente adopera il termine "integrazione". Per il biennio 2008-2009 le risorse sono assolutamente insufficienti e questo emendamento punta semplicemente ad un lieve incremento a renderle meno virtuali; punta cioè a rendere la base per il rinnovo contrattuale per la specificità, non più di 200 ma di 400 milioni di euro. Colleghi del centro-sinistra, votate pure contro questo emendamento in automatico come avete fatto finora per tutto ciò che ha riguardato le Forze di polizia; avrete un ulteriore motivo per non presentarvi - come avete fatto finora - agli incontri programmati tra i parlamentari e le rappresentanze ed i sindacati delle Forze armate e delle Forze di polizia, perché chi di voi dovesse comparire in queste sedi dovrebbe giustificare - lo ripeto - in presenza di extra-gettito un bilancio di tasche vuote e di autovetture ferme e magari dovreste anche spiegare in queste sedi che il solo impegno che, sulla base del programma dell'Unione, avete preso nei confronti delle Forze di polizia e che state tentando disperatamente di rispettare è l'istituzione della Commissione di inchiesta sul G8.

presidente, non abuserò del tempo concesso, ma credo sia doveroso dichiarare il voto di Forza Italia a favore di questo emendamento per le ragioni esposte. Non possiamo essere vicini alle Forze dell'ordine solo a parole e solo con le commemorazioni, dobbiamo esserlo anche negli atti. Dare loro i mezzi per fare ciò che gli chiediamo ogni giorno di fare per proteggere la sicurezza dei cittadini è - credo - un dovere di ciascuno e, quando ci sono i «tesoretti» che vengono dilapidati per motivi di tutt'altra rilevanza, davvero bisognerebbe riuscire a trovare una parte per questa importantissima categoria. L'emendamento fa questo e per tale motivo voteremo

si è proceduto in modo un po' strano: si sono dispensate risorse a pioggia un po' dappertutto e ci si è dimenticati, proprio nel momento in cui la Nazione tutta soffre di un'offerta di sicurezza pari alle esigenze e alla domanda che continua ad emergere, delle Forze armate e dei Corpi di polizia. Avevamo già detto che non era possibile eliminare addirittura i limiti che si ponevano alle assunzioni per certe categorie, tra cui il Corpo forestale dello Stato, ma quelle risorse dovevano essere accantonate per essere destinate alle Forze dell'ordine, Esercito, Carabinieri e Polizia, proprio per poter offrire quello che oggi tutto il Paese chiede: maggiore sicurezza, maggiori controlli, poter dormire

che ha prodotto. Non ricordo da anni che la Polizia, un corpo sempre ligio, sempre inquadrato, sempre ossequioso, abbia rotto gli schemi e sia dovuta venire due volte a Roma a protestare contro il Governo. Non si può chiedere a questi ragazzi di andare a morire e dopo non ricordarsi di loro quando è ora di far vivere le loro famiglie, dandogli delle miserie che fra un po' ci manderanno o vi manderanno di ritorno. Le Forze armate e la Polizia si ricordano sempre e non solo quando c'è da celebrare una cerimonia o un funerale di Stato.

perché questa è la somma complessiva delle richieste corporative che i diversi settori della maggioranza hanno avanzato per assicurare il loro consenso alla finanziaria - non si siano trovate poche decine di milioni di euro per la sicurezza.

il numero di addetti che vengono indicati da assumere in tale struttura ha anche ricevuto nella finanziaria un mandato preciso per il recupero di una determinata somma di evasione. come se si fosse assunto qualcuno perché si recasse presso le imprese e i contribuenti a recuperare una somma esatta, precisa, senza conoscere la dimensione del fenomeno o se questa visione sussiste o meno.

allora, la filosofia di questa maggioranza: non si spendono soldi per difendere i cittadini che vengono uccisi nelle loro case dalla delinquenza extracomunitaria, se ne spendono moltissimi per mettere in difficoltà quel ceto medio e quel ceto di produttori i quali cercano di resistere all'ingiustizia fiscale utilizzando tutti gli strumenti a disposizione della legge; cittadini dei quali si dice e si scrive - per esempio nel bollettino dell'Agenzia delle entrate - che usano la legge per evadere il fisco.

tassare le aziende indebitate ed eliminare l'indebitamento dalle deducibilità perché quello era un *escamotage* che le imprese avrebbero adottato per non pagare le tasse.

intervenire per motivare il voto contrario del Gruppo Forza Italia, soprattutto con riferimento al fatto che l'articolo 95 non contiene l'accantonamento per i rinnovi contrattuali. articolo, infatti, prevede per i rinnovi stessi un accantonamento pari allo 0,4 per cento del monte dei salari: si tratta di un incremento che corrisponde a quella che, nel gergo delle relazioni industriali, viene chiamata l'indennità carsica, cioè quella erogata nella presunzione della vacanza contrattuale. Invero credo che il Governo si accinga a non rinnovare i contratti, non avendo accantonato le risorse, o - cosa ancora peggiore a mantenere sommersa una grande voce di spesa, che mi permetto di considerare quasi obbligatoria. Mi sembra, infatti, obiettivamente difficile, nell'arco del biennio di riferimento 2008-2009, non procedere al rinnovo contrattuale. Secondo il minimo calcolo riferito all'inflazione programmata, nel biennio l'incremento dovrebbe essere del 3,2 per cento, pari a 4,2 miliardi

nel momento in cui, invece, la richiesta delle piattaforme contrattuali ovviamente include, oltre alla tutela del potere d'acquisto, anche incrementi legati alla produttività che noi auspichiamo non siano erogati a pioggia:

di risorse che costituisce un vero e proprio buco nei conti pubblici che dovrà necessariamente emergere, con i conseguenti problemi di copertura per dimensioni di questa straordinaria entità.

«Sentirsi dire, come mi è capitato questa mattina, dal Comandante dei Carabinieri che l'unico modo che ha trovato per fronteggiare le esigenze del servizio con le risorse disponibili è stato di dichiarare che la vita media delle automobili dell'Arma passa anni e mezzo a sei anni e fa la stessa cosa con gli elicotteri e che di conseguenza quello che dovrebbe essere speso per il rinnovo viene speso per le riparazioni e quello che dovrebbe essere speso per la manutenzione non è più disponibile, è certamente mortificante». Questo è quanto ha affermato il ministro dell'interno Amato prima del taglio di 280 milioni avvenuto con il cosiddetto decreto Bersani,

e dell'emigrazione. Si può discutere successivamente dove farlo, però le argomentazioni poste dal vice ministro Danieli non ci hanno convinto e il senatore Buttiglione ha ricordato le vicende e i ritardi conseguenti. L'altra questione concerne un'appostazione relativa alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, un modesto finanziamento per consentire alle delegazioni dei vari Ministeri di partecipare attivamente alla fase ascendente del processo d'integrazione europea. Assistiamo infatti ad un *deficit* di partecipazione da parte dei funzionari dei diversi Dicasteri che, quindi, non possono recepire quello che sta avvenendo in Europa. Credo che, considerate

parere contrario su tutti gli emendamenti, facendo rilevare che in Commissione abbiamo già approvato alcune modificazioni alle Tabelle, che riteniamo di confermare nel testo licenziato dalla Commissione. SARTOR, *sottosegretario di Stato per

senatore Buttiglione piccola cifra per permettere una grande riforma che consenta ad ogni Ministero di avere un nucleo di valutazione della fase ascendente della normativa europea, che segue poi anche la fase discendente di tale normativa, è un emendamento che risolve un problema fortemente sentito anche dall'attuale Ministro e dall'attuale Governo. Mi stupisco che il Governo si dichiari contrario ad una questione che sappiamo, anche per quanto è stato detto in Commissione, che sta a cuore perché è un elemento indispensabile di funzionalità della pubblica amministrazione nel suo rapporto con l'Unione Europea. Non lamentiamoci poi che siamo sempre gli ultimi nel recepimento delle direttive europee, se ci rifiutiamo di allocare le pochissime risorse che permetterebbero un efficiente funzionamento del

militare della NATO. Questo riconoscimento va apprezzato e salutato con grande piacere da questa nostra Assemblea, che gli augura tutto l'appoggio politico necessario per l'esercizio di questa funzione e gli formula i migliori auguri di buon lavoro.

confermo il grande interesse su questo emendamento, che propone una soluzione molto innovativa sulla destinazione degli utili delle fondazioni, ma, allo stato, il parere rimane contrario.

Inizialmente i proponenti sostenevano che si trattava solo di una proroga dal 2008 di un beneficio già esistente e che non fosse necessaria alcuna forma di copertura. Ora, di fatto, si tratta di un innalzamento di un sussidio già esistente, per cui è stato opportuno accantonare tale emendamento perché nella formulazione originaria determinava oneri privi di copertura. Quindi, la nuova formulazione consente di dare adeguata copertura a questa che è un'estensione dei benefici, non una semplice proroga al 2008. La proroga era già contenuta nel testo originario del disegno di legge finanziaria. Esprimo parere favorevole.

un'iniziativa della 9a Commissione permanente del Senato, tra l'altro votata all'unanimità all'interno del rapporto della Commissione stessa sulla pesca e sull'agricoltura, anticipa un utilizzo positivo di risorse già accantonate nella finanziaria precedente per l'IVA speciale per le attività di pesca e auspichiamo sia il primo passo di un'iniziativa ancora più robusta da accogliere e definire in sede di approvazione della finanziaria alla Camera dei deputati per quanto riguarda l'IVA in regime speciale e per quanto riguarda anche gli studi settore. Per questi motivi, esprimo il voto favorevole

*relatore*. Signor Presidente, abbiamo approfondito il tema con il Governo e le norme contenute in finanziaria di cui si chiede la soppressione costituiscono la traduzione

di questo emendamento, che è stato riscritto proprio nel tentativo di superare l'obiezione fatta in questo momento dal Governo.

concordato con il Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia, ma che vede sia il Consiglio comunale di Trieste, sia quello di Gorizia, cioè le zone interessate, totalmente contrarie. Per quanto riguarda il rilievo dell'Unione europea, se fosse così, dovrebbe essere inserita in finanziaria anche una norma che riguarda la Valle d'Aosta, evidentemente questa norma non è stata inserita perché la Valle d'Aosta sa che questa misura è importante per i cittadini e le imprese del suo territorio. Per quanto riguarda in particolare le zone di Trieste e Gorizia, voglio ricordare che questa realtà che nasce dall'immediato dopoguerra (per queste ragioni lo stesso presidente Andreotti ha voluto sottoscrivere questo emendamento), consente a queste nostre terre di combattere quella che in questo momento è una concorrenza sleale che ci fanno i Paesi vicini, in particolare la Slovenia. Come sappiamo, la Slovenia entra in Schengen alla fine di quest'anno, sarebbe un danno rilevantissimo per le aziende e per i nostri cittadini, pregherei quindi il Govrno ed il relatore di ripensare il loro atteggiamento anche a fronte di quello che ho detto e pregherei anche i colleghi della maggioranza, in modo particolare quelli che hanno sensibilità per le realtà

o rischiano sempre di vivere grossi pregiudizi. Pensiamo alla concorrenza che fa uno Stato frontaliero con le politiche fiscali ed economiche: certi prodotti in un Paese non si venderebbero assolutamente, ma si andrebbe ad acquistarli oltre confine. Ricordo all'indomani della guerra dei Balcani, la Slovenia si era staccata dalla ex Jugolsavia e praticava politiche di defiscalizzazione sui prodotti energetici e sugli idrocarburi

le famose fasce con prezzi decrescenti, anche per combattere, nell'interesse dell'economia nazionale italiana, questa concorrenza non sleale - perché non lo è - perché ogni Stato è libero, indipendente e sovrano di praticare le politiche che che ritiene. Per cui, è sicuramente da sostenere nell'interesse generale e nell'interesse di tutta la popolazione italiana, non solo di quella frontaliera e di Trieste.

Colleghi, ho preso atto che si è trattato di un errore da parte del collega Baldassarri, ma dal momento che il risultato è proclamato,

Esprimo apprezzamento e soddisfazione per l'accoglimento dell'emendamento che ha un valore, al di là del dato economico forse troppo limitato, importante dal punto di vista simbolico e dell'indirizzo politico. Riconoscere una detrazione importante dell'IRAP alle aziende che denunciano atti estorsivi utilizzando una norma della Regione siciliana e altre similari costituisce un'indicazione importantissima che aiuta un sentimento e un indirizzo forte che si sta diffondendo nella mia Regione e in altre nell'ambito dell'imprenditoria che comincia a denunciare le estorsioni. In un momento in cui la lotta alla mafia segna importanti risultati positivi, cominciare a compromettere quella base economica forte che deriva dalle estorsioni significa destabilizzare la potenza intimidatrice della mafia. Dovremmo ulteriormente sviluppare questo indirizzo rendendo conveniente la denuncia dei fatti estorsivi e innestando un processo virtuoso. Quindi, è una buona cosa che abbiamo fatto insieme.

Il Gruppo di Forza Italia sosterrà questo emendamento perché in un momento difficile in cui gli imprenditori siciliani stanno denunciando apertamente i loro estorsori e Confindustria ha fissato un codice di comportamento per cui chi sbaglia viene espunto dal sistema delle imprese, in un momento nel quale a causa delle ristrettezze economiche non è possibile garantire e presidiare bene il territorio con le forze dell'ordine alle quali spesso manca finanche la benzina per andare in giro con le volanti della Polizia di Stato, dare una detrazione fiscale a chi ha il coraggio di denunziare questo cancro terribile della mafia, che oltre che uccidere gli uomini uccide tutte le loro libertà e uccide la libera concorrenza, è un gesto del Parlamento di sensibilità verso la lotta alla criminalità organizzata che sembra non essere più nell'agenda politica di questo Governo.

condividendo peraltro pienamente un'idea sulla quale da tempo rifletto e scrivo, quella cioè che occorrerà fare in modo che si introducano leve positive per suscitare comportamenti virtuosi. spesso, la punizione minacciata e non eseguita è capace di prevenire comportamenti gravi e non sempre soccorre di fronte alla paura e alla soggezione. prevedere un premio, che lo Stato tessa un patto con le aziende che si rifiutano di sottostare al pizzo, è segnale di una attenzione grande che lo Stato ha nei confronti di questi comportamenti virtuosi. Nessuno ha mai pensato che la mafia, così come altri fenomeni criminali che hanno afflitto il nostro Paese in passato, possa essere sconfitta esclusivamente dalle forze di polizia o dentro le aule dei tribunali. Crediamo che sia assolutamente essenziale cominciare da qui e andare avanti sulla strada di un patto che premi i comportamenti virtuosi, li enfatizzi e faccia diventare, lasciatemi usare questa parola, conveniente essere contro gli interessi della mafia. Io ringrazio il senatore Pistorio per la presentazione di questo emendamento. Non so se i colleghi degli altri Gruppi che hanno sottoscritto l'emendamento vorranno prendere la parola, lo trovo un felice esempio di sintesi su una questione essenziale per il Mezzogiorno ma più complessivamente per il nostro Paese.

a favore di questo emendamento del collega Pistorio e lo farà convintamente perché come ben diceva la collega Finocchiaro introduce, grazie a questa normativa messa in pratica nella Regione siciliana, siciliana, un atteggiamento, una valutazione positiva, uno stare accanto a coloro che scelgono di stare contro la mafia e contro tutte le mafie. Noi riteniamo che questo sia importante perché apre un capitolo nuovo nel comportamento delle istituzioni, non soltanto repressivo ma attivo, di sostegno. Stare accanto a chi soffre tutte le aggressioni e tutte le ingiustizie è un fatto che sicuramente accende la speranza e suscita comportamenti positivi. Noi riteniamo che questo atteggiamento debba essere esteso a tutti quegli episodi di violenza sistematica, a tutti quei comportamenti che di fatto dimostrano di vedere nello Stato, soprattutto nello Stato che rappresenta il senso della nazione, un nemico. Ecco, quindi, una linea da seguire contro la mafia ma anche contro il terrorismo. Un comportamento importante che se le istituzioni riusciranno ad estendere a 360 gradi, certamente servirà a tenere sempre più vivo il senso dell'identità nazionale e a scoprirsi tutti impegnati in una battaglia a sostegno, soprattutto, del senso dello Stato.

Signor Presidente, annuncio il voto favorevole, tra l'altro già testimoniato dalla firma del Capogruppo di Sinistra Democratica,

in Sicilia, sia con riferimento alle azioni di questi giorni delle forze dell'ordine (che hanno assicurato alla giustizia coloro che si erano resi

e Impastato, senza l'intreccio con l'amministrazione, con le strutture economiche e con la politica non c'è mafia, non c'è il fenomeno della mafia in quanto tale. Perché la mafia è profitto, è beni, è percorsi di accumulazione, è percorsi di valorizzazione del capitale, è intreccio - oggi - tra economia legale e illegale, è borghesia mafiosa. Si devono allora aprire, anche grazie all'azione dello Stato magari minima ma importante come quella che questo emendamento evoca,

Colgo l'occasione per dire che sul sequestro e la confisca dei beni mafiosi - altro terreno particolarmente importante - dobbiamo fare presto passi avanti. Colgo l'occasione anche per dire al Governo presente qui in Aula e al Ministro dell'economia che come ha richiesto ad ampissima maggioranza la Commissione antimafia - anche attraverso il presidente Forgione - qualche giorno fa, è importante che si sblocchi il tema dell'agenzia autonoma che possa valorizzare e ridestinare alla socializzazione i beni sequestrati e confiscati ai mafiosi.

per la lotta alla mafia venga dalla Casa delle Libertà. Colleghi, vorrei ricordarvi che con grande innovazione in questa legislatura avete destinato per i fondi della Commissione antimafia, che dovrebbe operare contro la mafia per scoprirne tutte le intersecazioni con la società, il suo modo di operare e delinquere, 300.000 euro all'anno. Avete voluto fare le nozze con i fichi secchi mettendo la Commissione antimafia in condizioni di non operare: operare: è un peccato originale che vi portate addosso in questa legislatura. Questo non va mai dimenticato e io non cesserò mai di ricordarvelo, perché avete costruito una Commissione antimafia che non può operare, questo è il punto che va sottolineato. Non posso, però, neanche sottacere due questioni che mi lasciano un po' di amaro in bocca. La prima è che

gli stranieri in Padania hanno ammazzato, torturato, stuprato innumerevoli persone, (anche ieri è stato ucciso un medico a Milano) esce un trafiletto, si sente qualche espressione di cordoglio e basta; viene negli stessi termini massacrata una persona a Roma e si emana un decreto. Ecco, vorrei che questo doppiopesismo finisse una volta per tutte, perché noi abbiamo gravissimi problemi di ordine pubblico dalle nostre parti. Per favore, tenetene conto.

dell'emendamento, che considero umiliante per la Sicilia, al di là della buona volontà del senatore Pistorio e di chi ha sottoscritto una elemosina di 5 milioni di euro parcellizzata per tutti coloro che subiscono danni ed estorsioni si riduce al nulla.

Il Governo Prodi e la sua maggioranza hanno votato contro l'aumento della dotazione per le forze di polizia. Il Governo Prodi ha buttato a mare centinaia di milioni di euro per assumere dei precari lasciando a terra giovani che potevano partecipare e vincere concorsi, trasformandoli in potenziali disperati o forse anche delinquenti in futuro. Questa è la politica del Governo Prodi, che a me non soddisfa

Signor Presidente, onorevoli colleghi, desidero esprimere apprezzamento per l'iniziativa legislativa del senatore Pistorio, che ha felicemente compreso le ragioni di una sfida che sta dentro la realtà siciliana, con il suo carico di angosce e di sofferenze. Esse hanno trovato in questo emendamento un punto alto di risposta, anche se parziale, collocando felicemente l'azione del Governo nazionale nel solco della migliore tradizione per combattere la malavita organizzata e le mafie di ogni tipo, per costruire anche in Sicilia, e non solo, una rete di protezione a sostegno dell'imprenditoria sana. Auspico che ciò segni il tempo di una nuova primavera, di una stagione di attenzione vera dello Stato, di percorsi legislativi che camminino di pari passo con le potenzialità e le attese di un popolo massacrato dal devastante flagello della criminalità mafiosa.

e che deve portare le forze politiche di maggioranza e di opposizione a coniugare una nuova risposta dello Stato rispetto a questi *raid* che, giorno per giorno, massacrano la parte sana del Paese e ciò che di sano c'è nel mondo dell'economia e della finanza.

con cui il Senato vuole dare rilievo a una presa di posizione utile ed indispensabile, di cui si richiederebbe più spesso una sottolineatura nelle Aule parlamentari. Noi vorremmo che che si facesse a meno - lo dico garbatamente al senatore Castelli - di individuare le motivazioni che hanno portato il senatore Pistorio a Non è così

ha voluto assumere con grande forza la presa di posizione che l'ha caratterizzata, nel momento in cui il Presidente di Confindustria di Agrigento è costretto a muoversi con la scorta

la sottoscrizione da parte del Capogruppo vale implicitamente per tutti i componenti del Gruppo. Noi voteremo convinti. Sembra anche a me che quanto sottolineato dal senatore Castelli circa l'esigenza che misure di lotta debbano essere prese non solo relativamente alla Sicilia, e indipendentemente dal giudizio sulla quantità del valore economico della misura che prendiamo, sarebbe un atto opportuno sia da parte del Parlamento che del Governo.

Strano che è già intervenuto in dissenso dalla posizione ufficiale espressa dal collega Nania. PRESIDENTE. A questo punto, inverto l'onere della prova: chi volesse non sottoscrivere l'emendamento, lo segnali alla Presidenza.

che l'Assemblea si unifichi simbolicamente su questi emendamenti, al di là delle appartenenze di schieramento. Signor Presidente,

che per il contrasto alla criminalità organizzata, sia quella mafiosa sia quella più articolata che fa parte di altre tipologie di criminalità, la politica debba essere unita Il contrasto alla mafia non può essere appartenenza e patrocinio soltanto di una forza politica: questo è quanto vuole la mafia, cioè la divisione della politica, per inserirsi come il coltello nel burro nelle istituzioni e fare da padrone.

Occorre dare un segnale a chi è sottoposto a questa terribile criminalità, a chi vede la propria famiglia e la propria attività commerciale (spesso piccola e di carattere artigianale)

Presidente, credo che si debba dibattere su argomenti delicati come quello della *class action* e quelli riferiti all'articolo 91,

so che è in corso una procedura di applicazione di quanto previsto dall'ultima legge finanziaria. L'ordine del giorno deve servire per il prosieguo di tale operazione.

mediante l'istituzione di mercati in spazi aperti, destinati alla vendita solo da parte di agricoltori in forma singola e associata,

l'intervento al 2008, mantenendo lo stesso importo di 180 milioni di euro, poiché la copertura allo stato non è pienamente soddisfacente. Invitiamo quindi ad approvare questo emendamento, con parere favorevole subordinatamente all'approvazione del subemendamento, poiché la copertura dell'emendamento principale è decennale e quindi difficilmente sostenibile in questa fase. a seguito di questa approvazione, è necessario che il Governo in prosieguo, conformemente a quanto contenuto nell'ordine del giorno approvato da tutti, provveda ad individuare una copertura più idonea.

la disponibilità concreta di quanti hanno creduto, recepito e sostenuto la loro legittima richiesta. Essi vedranno soprattutto le istituzioni, in quanto tali, che rispondono in maniera positiva a queste richieste. Siamo fiduciosi, lo dico al ministro Turco e a tutti noi, che continueremo su questo percorso. É un percorso, e vorrei ricordarlo

è tangibile e, in divenire, è una cosa ottima. Colgo l'occasione, e concludo, per dire che talvolta la tanto bistrattata politica trova unità vera:

perché è un elemento fondamentale che ci consente oggi di rivedere i livelli essenziali di assistenza e quindi anche l'assistenza nei confronti di questi soggetti. Auspicavamo allora l'approvazione sia dell'abrogazione dei *ticket* che di un emendamento che intervenisse su tale questione; siamo soddisfatti che questo sia avvenuto già con il decreto sul 2007.

Il collega Massidda ha i tempi a disposizione perché non appartiene al Gruppo di Forza Italia.

Io sono parzialmente soddisfatto: passando da zero a 180 milioni, sarei ingiusto se non avessi un minimo di soddisfazione. Credo però di non essere stato mai ascoltato sufficientemente per spiegare ai tanti amici, che pensano di avere trovato la bacchetta magica, che uno stanziamento solo per un anno non risolve il problema alla stragrande maggioranza di queste persone. per il semplice motivo che non credo ci sia in Italia qualcuno che rinunci ad una transazione in nome di un'anticipazione senza avere la sicurezza di essere risarcito del tutto. Stiamo parlando ancora di una piccola frazione di una cifra molto più ingente che noi abbiamo chiesto di distribuire nell'arco di dieci anni. Questo Governo, che l'anno scorso aveva fatto il giro dell'Italia promettendo una soluzione ma non aveva stanziato un euro,

Ecco perché chiedo che ci sia qualcosa di più. Chiedo anche che sia supportata la Ministra, che qualche volta si è offesa e ha detto: non avete fiducia in noi. Ma come possiamo avere fiducia, non in lei, ma nel suo Governo, che ha promesso tanto e oggi dà una risposta parzialissima, suonando le campane a festa come se avesse risolto il problema per sempre? Ecco perché chiedo, lo ripeto, anche agli amici che hanno espresso grande soddisfazione,

per colpa dello Stato. Esse hanno avuto trasfusioni con sangue infetto non solo per colpa della malasanità ma proprio per le scelte scellerate di una sanità del passato troppo spesso governata dalle stesse persone che dall'altra parte, oggi, puntano il dito verso il centro-destra. *(Applausi dai

saputo fare. Però, a onor del vero, una piccola ricostruzione della verità: siamo arrivati qui, con il decreto, a chiedere giustizia, che venisse dato o risarcito, che lo Stato onorasse un obbligo morale ancora prima che giuridico, e il Governo ha detto di no. L'Assemblea ha obbligato il Ministro a rimangiarsi quel no, riconoscendo certi diritti a queste persone danneggiate loro malgrado. La seconda volta, in questa sede, il Governo ha detto no per l'ennesima volta ed è stata la grande insistenza dell'Assemblea, con

quasi graziati da questa piccola risoluzione, contenuta nell'emendamento del relatore, a noi sinceramente non piace. Ci dispiace moltissimo, invece, che abbiamo perso un'ottima occasione per continuare nella strada intrapresa attraverso il decreto legislativo. Ci era stato detto che avremmo trovato una soluzione in questa finanziaria, che sta passando dal Senato alla Camera. Ci viene ora detto che probabilmente la copertura verrà trovata alla Camera. il provvedimento tornerà al Senato blindato. Non so quale finanziaria dovremo aspettare per trovare la soluzione completa a questo problema.

Presidente, non credo che cinque minuti di discussione compromettano il soddisfacimento dei diritti. Le chiedo di restare nella sua funzione; si chiede

per mia colpa, ero distratto e non sono intervenuto nel dibattito. Vorrei precisare che il Gruppo di Alleanza Nazionale è favorevole a riprendere i lavori alle ore 15. Se c'è questa possibilità, saremmo lieti di poterne

i due minuti in più e mi sembra che negli interventi di oggi non vi sia stato alcunché di ostruzionistico, al punto che anche da parte della maggioranza